Ove necessario, i lavori potranno proseguire anche nella mattinata di venerdì 11. Domani, alle ore 16, il Ministro dell'interno renderà un'informativa sui fatti occorsi in occasione di recenti manifestazioni di studenti

che si terrà in Aula alle ore 16. La discussione del decreto-legge proroga stato di emergenza potrà eventualmente proseguire nella settimana dal 15 al 17 febbraio. Nella settimana dal 22 al 24 febbraio sarà discusso il decreto-legge proroga termini attualmente all'esame della Camera dei deputati. Giovedì 17 e giovedì 24 febbraio, alle ore 15, avrà luogo il *question time*. La Conferenza dei Capigruppo è peraltro nuovamente convocata oggi alle ore 17,30.

da lei citato. È iniziata la fase di illustrazione e di esame degli emendamenti, che sono 300; avevamo oggi la scadenza per presentare subemendamenti ad un emendamento del Governo molto corposo. Ritengo che per concludere i lavori in Commissione sia necessaria tutta la giornata di domani.

Signor Presidente, sabato 29 gennaio Ginevra Sorressa, una bambina di due anni di Mesoraca, nel Crotonese, è deceduta all'ospedale Bambino Gesù di Roma. La piccola, che, dopo essere risultata positiva al Covid un paio di giorni prima, aveva ricevuto le prime cure dai sanitari del 118 di Campizzi, è stata poi trasportata all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro già in condizioni critiche per la grave insufficienza respiratoria e da lì, con un volo militare, poiché bisognosa della ventilazione in ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation), all'ospedale pediatrico della Capitale, dove però le sue condizioni hanno reso vano l'intervento dei sanitari. Di norma, tragiche vicende come questa risvegliano solo per qualche giorno l'attenzione sulle carenze sanitarie che i calabresi affrontano quotidianamente a riflettori spenti. Nel territorio d'origine della piccola Ginevra in particolare, l'Alto Marchesato di Crotone, che comprende, oltre Mesoraca, Cotronei, Petilia Policastro, Santa Severina e Roccabernarda, l'utenza di oltre 26.000 residenti sta vedendo smantellare il proprio diritto alla salute. L'unico presidio sanitario è infatti un poliambulatorio negli anni progressivamente depotenziato, carente di personale e con gravi criticità strutturali, avviato a un'inesorabile chiusura nell'indifferenza della politica regionale, nonostante la costante mobilitazione dei cittadini. Dalle dichiarazioni dei sanitari di Catanzaro che l'hanno presa in carico, sembra sia stata fatale alla piccola Ginevra la mancanza in Calabria di un centro con terapia ECMO pediatrica, ma subito il presidente Occhiuto ha annunciato la creazione di una unità operativa complessa di pediatria a Catanzaro presso l'azienda ospedaliera universitaria. Da calabrese, pur augurandomi che quell'annuncio si concretizzi al più presto, vorrei invitare i responsabili della sanità regionale ad attuare ogni sforzo per affrontare integralmente la difficile situazione sanitaria di tutto il territorio, legata anche ma non solo alla carenza di personale medico che diserta costantemente i bandi regionali, chiamato in causa anche da Occhiuto nelle dichiarazioni ai *media.* Occorre una reale volontà di intervenire per creare condizioni migliori in termini di meritocrazia, implementazione tecnologica e digitale, possibilità di aggiornamento professionale continuo, per poter davvero attrarre i professionisti del settore sanitario in Calabria e avviare una svolta. In mancanza di competenze e capitale umano, invece, risulterebbe vano qualunque sforzo fatto in altre direzioni, dalla realizzazione di nuove strutture all'acquisto dell'apparecchiatura più moderna. In attesa di questa generale riorganizzazione, auspico che il presidente Occhiuto colga l'occasione per ascoltare finalmente il grido di aiuto della comunità alla quale apparteneva la bimba, ripristinando urgentemente i servizi essenziali di cui è stata privata. Sarebbe forse una tardiva forma di risarcimento morale a lei e a quei cittadini da troppo tempo trattati come figli di una Costituzione minore.

Si tratta certamente di un detenuto dal *curriculum* malavitoso di un certo spessore, ma che al momento versa in condizioni di salute davvero penose e aggravate dall'età di ottantotto anni. Oggi ho dunque l'occasione di focalizzare l'attenzione ancora una volta sulla condizione carceraria italiana, cioè il segmento finale di tutta la filiera giudiziaria in cui tutti i mali del Paese fanno capolino, salvo poi rimanere irrisolti in quei luoghi. È intollerabile che tutto ciò che non funziona debba rimanere a carico della polizia penitenziaria e degli operatori che vi lavorano,

non può più essere trascurata: urge mettervi mano e al più presto. Ad esempio, le misure alternative più volte ventilate non sono mai state attuate in modo sistematico, come questo caso meriterebbe, proprio per il rispetto della dignità della persona, che resta tale anche se detenuta. Nel discorso tenuto qualche giorno fa dal Presidente della Repubblica, è stato particolarmente incisivo l'appello che ha rivolto a noi parlamentari nel cercare soluzioni innovative. Non lasciamoci sfuggire questa occasione per compiere questa svolta epocale; si è trattato di un invito a tutti noi a trovare soluzioni più dignitose per quest'ampia categoria di persone che è la popolazione carceraria, la quale comunque non cessa di essere cittadina di uno Stato democratico.

questo mio intervento oggi fa parte di quell'iniziativa, voluta dalle donne del Parlamento, che abbiamo chiamato staffetta per le donne in Afghanistan. Il mio intervento dà voce alle donne e ai rifugiati che sono in Italia, che mi hanno pregato di essere la loro voce e di dire le loro parole. Quindi io parlerò a nome dell'associazione A2030. La situazione delle donne in Afghanistan sta peggiorando, non solo per il freddo, la crisi economica e la lotta per un pezzo di pane. Sul fronte dei diritti umani e civili si intensificano le persecuzioni delle giovani attiviste che si sono pubblicamente esposte nelle manifestazioni più recenti già inserite nelle liste nere per il loro operato negli anni della cooperazione con organizzazioni straniere. Le recenti notizie relative alla cattura e scomparsa di Alia Azizi, direttrice del carcere femminile di Herat, e delle altre ragazze attiviste catturate nei giorni scorsi fanno temere il peggio per le donne che hanno rivestito ruoli di rilievo quali giudici, avvocatesse, poliziotte, giornaliste e attiviste per i diritti umani. Allo stesso modo sono in pericolo tutte le studentesse, che formalmente hanno ancora diritto all'istruzione, ma che di fatto vedono chiusi i loro corsi di studio e chiedono il diritto di accesso all'istruzione. Saranno tollerati corsi di studio ritenuti adatti alle donne, invalidando percorsi di studio su cui le studentesse hanno investito anni e fatiche, ma soprattutto in cui avevano riposto le loro speranze. Alcune testimonianze raccolte dal progetto Afghanistan 2030-Next Leaders, promosso da Cultura Italia e dall'organizzazione di volontariato A2030, offrono un importante spaccato di questa realtà, su cui possiamo e dobbiamo agire, in Italia, per le giovani donne pronte a ricominciare una nuova vita, e in Afghanistan, per le donne ancora in pericolo. Tra le poche fortunate che sono riuscite a lasciare il Paese abbiamo accolto in Italia: laureata in infermieristica con tre anni di esperienza nel dipartimento vaccinazioni, che spera di poter proseguire la sua carriera in Italia; docente di informatica, esperta di linguaggio Java; informatica ricercatrice, che ha sviluppato uno studio; laureata in economia e studentessa del *master* in scienze economiche. E molte altre, delle quali purtroppo non possiamo fare il nome. Con Afghanistan 2030-Next Leaders si sono individuate cinque differenti strategie di intervento, a seconda del *target* dei destinatari: studentesse, attiviste, docenti, professioniste e imprenditrici. Questo è un progetto importante, caratterizzato da una progettazione partecipata con i beneficiari degli interventi, sviluppando le loro richieste di intervento su temi e *target* ritenuti prioritari e sviluppando una rete di partenariato agevoli il *matching* tra i profili selezionati e le opportunità di inserimento socio-economico, con il coinvolgimento del settore privato. Per le studentesse e gli studenti che intendono proseguire gli studi si intercettino opportunità di borse di studio sostenendo i candidati nel percorso di selezione, immatricolazione e trasferimento territoriale, anche grazie al supporto di Refugee Welcome Italia. Per i docenti si avviino i contatti con gli atenei accoglienti, indicando l'opportunità di borse di ricerca e posizioni di *visiting professor*. Per le professioniste e le imprenditrici sia attivata una collaborazione con Migrants, per la validazione delle competenze pregresse (è importante questo) e per il *matching* con il mercato del lavoro; un accompagnamento all'imprenditoria migrante. Sul fronte internazionale stiamo sostenendo studentesse e docenti titolari di borse di studio in Italia, ma le condizioni di ottenimento del visto non sono assolutamente favorevoli. L'attivazione di programmi di imprenditoria che abbiano come modello il commercio equo e solidale e di corsi universitari *online* sono tra gli obiettivi più ambiziosi che si vorrebbero realizzare. Per i profili più qualificati sarebbe inoltre possibile inviare aiuti attraverso il programma di Migrants e attivare dei corridoi di ingresso protetti attraverso il *matching* lavorativo con aziende ricercanti specifiche competenze. I primi riscontri lasciano presagire che la strada intrapresa è quella giusta, tuttavia serve ancora un appello alle istituzioni. Ci sono persone bloccate da mesi in Pakistan: ad esempio

era nelle liste di espatrio già ad agosto e oggi vive nascosta in un rifugio a Kabul, dove a breve metterà al mondo suo figlio senza poter lasciare il suo nascondiglio.

un appello anche alle confederazioni professionali affinché promuovano opportunità di inserimento qualificato, *internship* e opportunità di formazione e conversione dei titoli, ad esempio per le donne avvocato, giornaliste e attiviste dei diritti umani che sono ancora a Kabul. Serve che i canali di aiuto della politica internazionale eleggano canali femminili di distribuzione degli aiuti. Siamo qui per portare la testimonianza di quest'associazione di donne che sono in Italia, ma che ci chiedono aiuto. *(Applausi)*.